La seduta è aperta

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Presidente, scusate la voce, ma purtroppo mi è andata via. Onorevole Ministro, il mio quesito acquista oggi un significato - secondo me - ancora più importante e imponente, perché cade nel giorno dell'Europa e della pace, nel Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e in un periodo in cui purtroppo vi è il tentativo coattivo - da lei per fortuna fortemente stigmatizzato - di arruolare giovani italiani, francesi ed europei, per delle guerre che sono purtroppo in corso. In Italia si era persa la memoria - come avvenne avvenne per la tragedia delle foibe, dove morirono circa 5.000 italiani - del dramma e del destino dei cosiddetti legionari italiani, perlopiù altoatesini, della mia terra, ma anche giovani strappati alle zone depresse del Piemonte, del Friuli, della Sicilia e dell'Abruzzo, che furono arruolati in maniera subdola con una campagna manifesti

un addestramento atroce, del quale quei ragazzi non sapevano niente. È una storia tornata alla memoria in questi giorni semplicemente grazie ad un giornalista altoatesino, Luca Fregona, che ha scritto due libri editi dalla casa editrice altoatesina Athesia di un noto ex parlamentare,

della Legione straniera, attestata dal Bureau des anciens de la Légion étrangère, che la scheda di Alfredo Decarli avrebbe comportato il conferimento della Croce di guerra per i teatri di operazione esteri con la stella d'argento. Alfredo Decarli è partito per l'Indocina in cerca di uno stipendio per poter sposare la sua ragazza. È quasi una trama hollywoodiana. Come lui lo hanno fatto altre centinaia di migliaia di nostri ragazzi; erano circa 10.000 quelli che son stati arruolati dalla Legione francese in Italia e circa 1.300-1.500 sono morti a Dien Bien Phu. Ecco, Ministro, le chiedo se l'Italia si vuole mettere una mano sul cuore e chiedere ovviamente alla Francia non solo di restituire un luogo dove poter piangere i nostri ragazzi morti in quella guerra che non apparteneva loro, ma soprattutto che vengano loro riconosciute le pensioni di guerra. Alfredo Decarli, infatti, come tanti altri, ha consacrato la sua vita per una Nazione che non era la sua e non ha visto riconosciutagli la stella d'argento. Signor Presidente, desidero ringraziare la senatrice Biancofiore per aver posto l'attenzione sul tema dei cittadini italiani arruolati nella Legione straniera francese e caduti durante la guerra d'Indocina, soprattutto nella battaglia di Dien un dramma che ha riguardato migliaia di famiglie italiane, soprattutto della Regione Trentino-Alto Adige. Nella gran parte dei casi si trattava di migranti economici che hanno lasciato il nostro Paese, uscito dalle macerie della Seconda guerra mondiale, alla ricerca di un lavoro e di migliori condizioni di vita. Giovani italiani che sono poi rimasti coinvolti nella tragica campagna militare francese in Indocina, culminata nella sconfitta di Dien Bien Phu, dove molti di loro, come dicevamo, hanno perso la vita. Proprio due giorni fa è caduto il settantesimo anniversario di quella sanguinosa battaglia. Considero doveroso da parte del Governo tenere viva la memoria di questa dolorosa vicenda e per questo ho chiesto alla nostra ambasciata a Parigi di farsi parte attiva con le autorità competenti francesi al fine di acquisire informazioni sul caso del connazionale Alfredo Decarli e degli altri italiani caduti nella legione straniera In particolare, nel dialogo con le autorità francesi, verrà attirata l'attenzione sull'eventuale mancata corresponsione di indennità o altri riconoscimenti previsti dalla legge francese. È una vicenda umana dolorosa che il Governo continuerà a seguire con attenzione e vicinanza e, onorevole senatrice, appena avremo risposte concrete, le faremo sapere cosa ci dicono le autorità francesi.

L'unica cosa che mi permetto di sottolineare è che questi ragazzi non erano giovani migranti, almeno non quelli altoatesini. Erano proprio adescati casa per casa; addirittura ci sono sui giornali altoatesini dell'epoca le denunce fatte dai genitori rispetto al fatto che c'erano degli adescatori pagati dalla Francia. Il patto era chiaro: tu combatti per per la Francia, la Francia ti dà un buono stipendio, vitto, alloggio e, al congedo, anche un lavoro e la cittadinanza, patto - anche questo - che è stato disatteso. Confidiamo molto in lei, onorevole Ministro, perché oggettivamente queste famiglie hanno bisogno di giustizia, di poter piangere dei corpi e anche ricevere le relative indennità.

Signora Presidente, signor Ministro, la mia interrogazione e quelle che seguiranno riguardano il caso di Matteo Falcinelli, un nostro giovane connazionale che tra il 24 e il 25 febbraio è stato protagonista di una orrenda avventura.

avrebbero chiamato la polizia per mediare, diciamo così, e in realtà la cosa si è poi risolta in un'orribile scena che non possiamo che definire di tortura. Il povero Falcinelli è stato prima trattato con quella pratica che viene chiamata *hog-tie*; tutti la conoscono perché è stata la causa della morte di George Floyd, cioè il ginocchio posto sul collo della persona fermata che impedisce di respirare; poi ancora peggio, quando è stato portato nel commissariato, è stato letteralmente incaprettato, è stato cioè legato in modo tale che braccia e gambe fossero collegate, messo a pancia sotto in una posizione nella quale diventa difficile respirare, ed è stato lasciato lì in quelle condizioni per circa un quarto d'ora. Oggi tra l'altro è uscito un ulteriore viene detto a Falcinelli ammanettato: stai buono perché altrimenti potresti passare dei guai peggiori. La mia domanda è molto semplice: tra il 24 e il 25 febbraio, quando tutto questo è successo, e il 4 e 5 maggio, quando questi video sono usciti, che cosa ha fatto la Farnesina nei confronti del Governo degli Stati Uniti? Guardi, a me non convince chi dice che l'Italia non può dare lezioni sui diritti umani, perché le nostre carceri e i nostri detenuti sono anche in condizioni difficili, perché secondo me - come giustamente ha scritto Luigi Manconi qualche giorno fa - si possono sempre dare delle lezioni, si devono dare delle lezioni, soprattutto ai Paesi amici alleati. E quando c'è un caso di tortura di un connazionale, di un trattamento inumano e degradante, bisogna far sentire forte la voce del nostro Governo. Così come, sottolineo, gli americani hanno fatto sentire la voce del loro Governo e della loro opinione pubblica, per esempio, nel caso degli assassini del carabiniere Cerciello Rega, uno dei quali fu fotografato bendato e ammanettato. L'opinione pubblica americana giustamente si ribellò, la CNN e il «The Washington Post» scrissero su questo tema, perché era un caso di trattamento inumano e degradante fatto in un Paese amico e alleato. Quindi la domanda è semplice:

praticamente, la famiglia su che cosa ha potuto contare da parte del Governo italiano, a parte la normale pratica consolare che si attua anche a Orlando, quando qualcuno viene arrestato per aver rubato qualcosa a Disneyworld?

ho detto pubblicamente, sono rimasto profondamente colpito dalla violenza e dal tipo di trattamento al quale è stato sottoposto il nostro giovane connazionale Matteo Falcinelli da parte della polizia di Miami. Con equilibrio e rispetto per le istituzioni statunitensi, ma con tutta la forza necessaria, ho seguito da subito il caso e continuerò a seguirne gli sviluppi. Non appena viste, sabato notte, le immagini di quanto è accaduto, già nella prima mattinata di domenica abbiamo sollevato la questione con l'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma. Abbiamo lamentato il trattamento riservato al nostro connazionale e chiesto di sollecitare la massima attenzione da parte delle autorità americane. Ho poi telefonato alla madre di Matteo Falcinelli per esprimere la nostra vicinanza e l'impegno a continuare a seguire la vicenda. La signora ha pubblicamente ringraziato il Governo e il console generale a Miami, che sin dall'inizio aveva seguito il caso e prestato assistenza alla famiglia per gli aspetti legali. Non appena appreso, tramite le immagini divulgate, dei trattamenti subiti dal giovane, il console generale ha presentato una nota di protesta ufficiale. La nota, indirizzata al Dipartimento di Stato e al capo della polizia di Miami, ha evidenziato l'inaccettabilità di quanto accaduto. Il console generale vedrà proprio oggi il capo della polizia. Ieri il portavoce del Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che il Governo federale, dopo l'intervento italiano, riconosce le preoccupazioni sollevate sollevate da noi e dalla famiglia sulle circostanze dell'arresto di Matteo. Ha aggiunto che la polizia di Miami ha aperto un'indagine interna sul caso e che lo stesso Dipartimento di Stato continuerà a monitorare la vicenda. È uno sviluppo importante, frutto della nostra azione a tutela del diritto del nostro connazionale. Ho accolto con soddisfazione queste dichiarazioni, perché il Governo federale ha risposto prontamente e positivamente a una nostra richiesta di chiarimenti. Il nostro Governo continuerà a seguire il caso con la massima attenzione; io stesso incontrerò la prossima settimana alla Farnesina l'avvocato incaricato dalla famiglia di seguire la vicenda.

nella notte tra il 4 e 5 maggio, ma quei video risalgono al 24 e 25 febbraio. Noi abbiamo visto il ragazzo escoriato, ma lui ha denunciato subito le cose che erano successe. Purtroppo, questo caso assomiglia molto, per esempio, a quello di Ilaria Salis e a quello di Filippo Mosca, dove lei si muove sempre quando il caso tocca già le pagine dei giornali e diventa un caso allarmante, ma io so per esperienza, avendo servito nel suo Ministero, che la rete diplomatica e consolare fa arrivare alla Farnesina le notizie molto prima e per questo io le ho chiesto cosa ha fatto nel frattempo. Anche col caso Salis, infatti, lei ha risposto all'interrogazione dicendo che noi abbiamo 2.500-2.600 italiani all'estero e li trattiamo tutti alla

Così lei si è mosso quando si è mossa tutta l'opinione pubblica italiana, ma che ce l'abbiamo a fare un Ministro degli affari esteri che si muove quando arrivano i giornali? Conoscendo la diplomazia Conoscendo la diplomazia italiana, sono sicuro che sulla sua scrivania arrivano le segnalazioni complete di tutti i dati: così è arrivata da Budapest, così è arrivata nel caso Mosca dalla Romania, così è arrivata anche in questo caso.

prima che venissero divulgate quelle terribili immagini. Non voglio ripetermi rispetto a quello che ha detto il collega Scalfarotto, ma vorrei vorrei sottolineare che l'incaprettamento al quale è stato sottoposto il nostro concittadino, ovvero l'immobilizzazione per lungo tempo mediante una tecnica che causa intenso dolore,

Magherini. Come Sinistra Italiana, oltre a manifestare la ferma condanna in tutte le sedi, come dovrebbe fare anche lei,

Io non ho interrotto nessuno, signor Presidente. È una questione di buona educazione e di rispetto degli altri, ma evidentemente non sono abituati a rispettare gli altri.

internazionale*. Anche i senatori devono essere educati. Essere senatore non significa che uno può fare quello che gli pare, perché ci sono delle regole.

della senatrice che ha posto l'interrogazione. Quindi adesso lasciamo al Ministro la possibilità di rispondere. Se la senatrice non vorrà replicare o invece replicherà lei, lo deciderete voi. Mentre sento che c'è insoddisfazione per la mia risposta, però sono molto soddisfatto per le dichiarazioni della signora Falcinelli, la mamma di Matteo, che ha ringraziato il Governo e ha ringraziato il consolato e per me quello che conta è l'apprezzamento della famiglia e non una valutazione di tipo politico. *(Applausi)*. Detto questo, non appena ho visto le immagini dell'arresto di Matteo Falcinelli, ho chiamato sua madre per offrire la mia più calorosa solidarietà e quella di tutto il Governo italiano. Ho confermato che il consolato generale di Miami e tutta la Farnesina continueranno a seguire il caso giudiziario e a fornire massimo sostegno al nostro connazionale. Dopo aver avuto la notizia dell'arresto, il console generale si è subito attivato per prestare ogni necessaria assistenza, in particolare alla madre del connazionale, nelle relazioni con le autorità e con il legale. Nei costanti contatti con la famiglia il consolato ha anche fornito nomi e recapiti di altri legali specializzati che potessero tutelare e assistere il connazionale nel prosieguo della vicenda giudiziaria. Come avete letto sulla stampa, ripeto, la famiglia ha molto apprezzato l'attenzione del Governo e ha ringraziato il Governo e il consolato per l'assistenza fornita sin dall'inizio. Continueremo a seguire la vicenda con la massima attenzione, anche grazie alla nuova unità della Farnesina per la tutela degli italiani all'estero, creata il 1° gennaio scorso. Il potenziamento della precedente struttura, da me voluto, testimonia l'attenzione che dedichiamo a ciascuno dei nostri connazionali all'estero; lo facciamo in un quadro di continuo e silenzioso lavoro che ci vede attivi in tutti i continenti. Come ho illustrato rispondendo al quesito precedente, abbiamo subito sollevato la questione e lamentato il trattamento riservato al nostro connazionale con l'ambasciata degli Stati Uniti a Roma. Il console generale d'Italia a Miami ha presentato, come ho detto, una nota di protesta ufficiale per sottolineare l'inaccettabilità dei trattamenti subiti dal giovane. Lo stesso console generale, ripeto, vedrà oggi il capo della polizia a Miami. La prossima settimana incontrerò alla Farnesina l'avvocato Francesco Maresca, legale incaricato dalla famiglia di Matteo Falcinelli, per valutare insieme la vicenda e fornirgli l'assistenza del Ministero per i prossimi passi.

Mi verrebbe da farla parlare con il papà di Ilaria Salis, ma sorvoliamo. Vorrei cogliere l'occasione per affrontare un argomento che mi è molto a cuore. Dobbiamo tener presente che, se si è venuti a conoscenza dei gravi atti di violenza commessi ai danni del nostro concittadino, è esclusivamente grazie alle cosiddette *bodycam*. Nel nostro Paese sappiamo bene che esse non vengono utilizzate o vengono utilizzate in maniera discrezionale.

comprendere la diffidenza che da questi banchi si ha nei confronti dell'operato del Governo, del suo Presidente del Consiglio e anche del titolare della Farnesina. Se dovessimo infatti parametrare il comportamento che noi pensiamo debba essere tenuto davanti a questa gravissima vicenda da parte del Governo sulla base di quello che

doverosamente molto preoccupati e diffidenti. La vicenda di cui il senatore Scalfarotto e la senatrice Cucchi hanno parlato non c'è bisogno che venga ulteriormente illustrata, ma è stata veramente barbara. Ancora di più lo è stata, perché avviene in uno Stato democratico che è storicamente la Patria dei diritti dell'uomo; avviene in uno Stato all'interno di un Paese nel quale negli ultimi vent'anni sono avvenuti una cinquantina di episodi di questo tipo che sono andati a volte oltre i limiti della tortura. È stata una cosa veramente barbara da fare nei confronti di un ragazzo. Intervengo su questo argomento anche perché si tratta di un mio corregionale. La comunità tutta, non solo in Italia, ma l'opinione pubblica europea e anche mondiale statunitense è rimasta scioccata da quei fatti, e tuttavia la comunità di Spoleto, la città dove è nato questo giovane, lo è rimasta ancora di più, perché tra l'altro conoscono

probabilmente in ritardo, in seguito alla sollecitazione della stampa e non prima, ma noi vogliamo davvero capire cosa fate per non lasciare sola la famiglia, la quale si aggrappa giustamente a ciò che può. Il ragazzo ha ricevuto anche minacce quella sera e non solo: gli è stato

poco cancellabili. Dunque noi chiediamo, oltre che far sentire davvero la vostra voce, la voce del Governo del Paese nei confronti degli Stati Uniti, cosa farete concretamente per assistere la famiglia legalmente e per dare un contributo quotidiano in questo difficile percorso?

innanzitutto per me conta non l'interpretazione della soddisfazione o meno della famiglia, meno della famiglia, ma quello che ha detto la famiglia, quello che ha detto la madre di Matteo Falcinelli, che ha ringraziato il Governo italiano, ha ringraziato il Ministro degli affari esteri, ha ringraziato il consolato italiano *(Applausi)* per ciò che è stato fatto Poi le interpretazioni politiche sono libere e legittime. Ognuno può dire ciò che vuole, siamo in democrazia, per fortuna, ma anche io posso dire quello che è, perché questi sono i fatti. se c'è un'interpretazione diversa delle parole, una esegesi delle parole della signora Falcinelli, questo è un altro discorso. La signora Falcinelli ha ringraziato il Governo e il consolato in tutte le trasmissioni televisive dove è stata. dove è stata. I fatti: Matteo è stato arrestato dalla polizia statunitense a Miami nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, accusato di una serie di reati, tra i quali resistenza non violenta a pubblico ufficiale. Il fermo sarebbe avvenuto all'esterno di un locale notturno dopo un alterco con le Forze di polizia. Falcinelli è stato dapprima portato per alcune ore presso il centro di detenzione del Dipartimento di polizia di Nord Miami Beach. Qui le autorità di polizia gli hanno riservato un trattamento particolarmente violento e lo hanno immobilizzato collegando le mani ammanettate ai piedi legati. Lo testimoniano le stesse videocamere dei poliziotti. In seguito Falcinelli è stato trasferito presso una struttura penitenziaria. Il 28 febbraio il connazionale è stato rilasciato su cauzione. Da allora si trova nel suo appartamento a Miami, assistito dalla madre. Da un punto di vista legale, lo scorso 26 aprile un capo di imputazione - l'accesso non autorizzato a proprietà privata - è stato stralciato. una nuova azione da parte della magistratura e questo prevede, dopo un periodo di buona condotta vigilata dai servizi sociali, la possibilità di non avere conseguenze sotto il profilo penale. Si tratta di uno sviluppo positivo. Lo strumento, infatti, è pensato per dare una seconda possibilità agli incensurati. Dopo aver raggiunto questo importante obiettivo, la famiglia ha contattato i media, diffondendo i video e rendendo noto il trattamento violento applicato a Matteo da parte della polizia, che altri non avevano. Il giovane ha detto di voler restare in Florida per terminare gli studi e poi cercare di inserirsi nel mondo del lavoro. Come illustrato rispondendo ai quesiti precedenti, il consolato generale sin dall'inizio ha seguito il caso e prestato assistenza alla famiglia per gli aspetti legali. Non appena appreso tramite le immagini divulgate del trattamento violento cui è stato sottoposto il connazionale durante la detenzione, lo ripeto, abbiamo protestato con l'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, con il Dipartimento di Stato e con il capo della polizia di Miami. Prontamente il Dipartimento di Stato ha risposto in maniera positiva alla nostra richiesta di chiarimenti. Le ripeto che, per quanto riguarda l'assistenza legale, l'altro ieri mi è arrivata una lettera da parte dell'avvocato incaricato l'altro giorno dalla famiglia, che ha lo studio legale a Firenze, un avvocato penalista presso il foro di Firenze, che mi ha chiesto di incontrarlo. Gli ho detto di vederci domani, ha detto che domani non può e gli ho fissato un appuntamento la prossima settimana. Quindi la tempestività c'è stata, comunque, e come sono sempre abituato a fare. Anche per quanto riguarda l'assistenza legale, le ripeto tutto ciò che stiamo facendo e che sto facendo personalmente con il suo avvocato, che è un penalista incaricato dalla famiglia, che lavora presso il foro di Firenze. Anche noi esprimiamo insoddisfazione, perché pensiamo che si debba fare di più. Per esempio, non sappiamo niente su cosa stia facendo il Governo per favorirne il ritorno in Italia, nel rispetto delle norme e delle leggi, naturalmente anche di quelle statunitensi, perché è importante che Matteo torni al più presto in

Non è un atto tanto per fare, di prammatica. È il minimo sindacale per la dignità del nostro Paese il rispetto dei diritti e della dignità dei propri concittadini, anche all'estero. Infine, lo si faccia davvero per Matteo Falcinelli e davvero noi vigileremo sull'operato suo e del Governo, ma lo si faccia per tutti coloro - li abbiamo citati e lo ripetiamo - i cui diritti sono trattati in maniera incredibilmente irrispettosa, lo si faccia per tutti i nostri connazionali, a partire a partire da Ilaria Salis, per la quale il Governo nei confronti del Governo di Orban non ha usato il rigore e la fermezza che avrebbe dovuto usare.

Sin dal lancio del Piano Mattei da parte del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, in occasione del vertice Italia-Africa del 28 e 29 gennaio 2024, il Governo italiano ha posto l'Africa al centro della sua azione di politica estera, tanto sul piano politico-securitario quanto su quello economico-commerciale. In questa cornice, la cabina di regia per l'internazionalizzazione dell'8 marzo scorso ha definito il Continente africano come area geografica paritaria nell'ambito dell'azione di sostegno pubblico all'*export* e all'internazionalizzazione del sistema economico italiano per il 2024, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione economica con il Continente, alimentando un circolo virtuoso di sviluppo e di crescita. A tal fine, nella mattinata di mercoledì 8 maggio si è tenuto, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il primo *forum* di dialogo imprenditoriale Italia-Africa, con la partecipazione di delegati africani e italiani delle rispettive comunità di affari. Si chiede di sapere, onorevole Ministro, quali saranno i seguiti dell'iniziativa illustrata e quali azioni intende intraprendere il Ministro in indirizzo per dare ulteriore impulso all'azione di sostegno all'*export* verso l'Africa

Presidente, l'Africa è al centro della nostra politica estera, a partire dalla Presidenza del G7, e ad esse ha voluto dedicare la sessione di apertura della riunione dei Ministri degli esteri a Capri, cui ha partecipato la Presidenza dell'Unione africana, rappresentata dal Ministro degli esteri della Mauritania. Intendiamo trovare soluzioni comuni alle sfide globali del nostro tempo e favorire la crescita dell'intero Continente. La prosperità condivisa è il miglior strumento per sviluppare un partenariato paritario e stabilizzare le aree di crisi. Ciò consente anche di fronteggiare l'immigrazione irregolare e contrastare l'odioso traffico di esseri umani. I nostri scambi commerciali con l'Africa nel 2023 hanno sfiorato i 60 miliardi di euro e gli investimenti superano i 26 miliardi. Vogliamo incrementare, questi numeri importanti e rendere le comunità imprenditoriali le vere protagoniste del Piano Mattei. Il 24 aprile ho presieduto a Palazzo Chigi la seconda riunione della cabina di regia. Il saper fare italiano può diventare una componente essenziale per lo sviluppo del Continente e la diversificazione della sua economia. Penso ad esempio alla trasformazione *in loco* delle materie prime, ma anche alla formazione. Abbiamo incrementato le borse di studio per i giovani africani, favorendo i canali di immigrazione legale. Investiamo nel trasferimento di conoscenze e nella valorizzazione del capitale umano, sostenendo la creazione di *joint venture* attraverso numerose iniziative. All'Africa abbiamo riservato 200 milioni di euro del fondo Simest per l'internazionalizzazione delle imprese. Stiamo lavorando al Business Forum, con incontri settoriali presentazioni Paese. Il Forum di dialogo imprenditoriale Italia-Africa, che per la prima volta ho voluto organizzare, ha visto ieri la partecipazione alla Farnesina di 140 delegati da 21 Paesi, in rappresentanza di 47 associazioni di categoria. Transizione energetica e digitale, mobilità sostenibile, meccanica strumentale e agroindustria sono i temi al centro della discussione, arricchita altresì da 150 incontri bilaterali tra imprese. Cassa depositi e prestiti ha firmato cinque protocolli d'intesa con le banche multilaterali di sviluppo presenti all'incontro, con l'obiettivo di favorire la partecipazione delle aziende italiane alle gare d'appalto internazionali nei Paesi africani. Italia e Africa condividono un destino comune e, di fatto, grandi sfide, ma anche enormi opportunità. Il Governo lavora per rendere il partenariato con l'Africa una realtà concreta del presente e una prospettiva solida e credibile per il futuro.

da una parte, un Mediterraneo e un'Africa luogo di scambi economici, commerciali, culturali, politici, luogo di incontro tra culture diverse, esempio per il mondo di incontro di civiltà; dall'altra, lo scontro di civiltà e la catastrofe. Mi pare anche chiaro che ci sia l'ambizione in questo Governo di indicare a buona a buona parte dell'Europa la strada per diminuire quell'enorme divario che ancora esiste tra il Nord e il Sud del mondo, che è la grande questione sociale della nostra epoca. Grazie davvero Ministro.

Signor Ministro, con il decreto ministeriale del 16 dicembre 2022 è stato istituito il sistema di qualità nazionale per il L'obiettivo è di valorizzare le aziende virtuose e, al contempo, fornire ai consumatori informazioni corrette sulle modalità di produzione, vista la crescente sensibilità al riguardo. Pur essendo un passo in avanti, il sistema è su base

che dovrebbe riferirsi alla provenienza, al metodo di allevamento, al luogo del macello e alla distanza percorsa dall'animale fino alla macellazione. Questo va a svantaggio di chi sceglie la strada dei piccoli circuiti di produzione e l'allevamento degli animali adeguato alla specie. Un sistema di etichettatura trasparente consentirebbe ai consumatori di acquistare carni di qualità e di disincentivare la produzione di carni da allevamenti intensivi trasportati per lunghe distanze, in condizioni spesso insopportabili per gli animali. Allo stesso tempo, sarebbe uno strumento a disposizione del Governo per indirizzare maggiori risorse verso quelle produzioni a ridotto impatto ambientale e rispettose del benessere animale; in pratica, quelle che ricorrono alle migliori pratiche zootecniche, compreso l'allevamento all'aperto e quello transumante, tipiche delle produzioni tradizionali e dei piccoli allevatori. Si chiede pertanto di sapere: qual è il numero complessivo di operatori che hanno aderito al Sistema di qualità nazionale zootecnia; in che modo i rivenditori finali promuovono le produzioni di qualità all'interno delle attività commerciali; quali sono i vantaggi complessivi da esso eventualmente derivati in termini di miglioramento del benessere animale e di impatto ambientale. le chiedo se non concordi sull'opportunità di introdurre un sistema di etichettatura univoco, trasparente e obbligatorio per tutte le produzioni, che riporti informazioni chiare e soprattutto in ordine alla provenienza, alla modalità di allevamento degli animali

acquistano e consumano e - dall'altra - a valorizzare il grande lavoro di qualità che fanno in Italia i nostri produttori e trasformatori, che hanno la capacità di rendere più sicuri e qualitativamente più elevati i loro prodotti. Ed è per questo che la trasparenza può servire ad aumentarne ancor di più il valore sui mercati nazionali e internazionali. Riteniamo sia fondamentale porre il cittadino nella condizione di poter compiere scelte informate su ciò che consuma e creare un approccio nuovo e consapevole che porti alla riduzione degli sprechi e alla valorizzazione dei prodotti di qualità. A dicembre 2023, congiuntamente al Ministero della salute e al Ministero delle imprese e del Made in Italy, abbiamo disposto la proroga per tutto il 2024 del regime sperimentale di etichettatura trasparente, che impone di indicare l'origine sulle carni suine trasformate, così come sull'origine delle materie prime per la pasta, il riso, il pomodoro, il latte e i prodotti lattiero-caseari. Voglio ricordare in proposito anche i quattro decreti adottati nel mese di aprile 2023, con con i quali è stata imposta l'indicazione chiara in etichetta della presenza di farine di insetti nella preparazione di prodotti alimentari, con un'ulteriore previsione normativa, che è quella di avere scaffali separati dagli altri prodotti, in modo tale che chi vuole consumare insetti si dirige verso quegli scaffali e chi invece ritiene sia per per lui inopportuno non corre il rischio di sbagliare. Per questa ragione, però, noi contrastiamo qualsiasi tipo di etichettatura condizionante non informativa, come il Nutri-score; non lo facciamo da oggi e non lo facciamo da soli, perché la maggior parte di questa assise ha condiviso la battaglia proposta da Fratelli d'Italia all'epoca con un ordine del giorno che pose l'allora Governo nella condizione di rafforzare l'impegno in Europa ed evitare che tale etichetta divenisse di uso comune. Il Sistema di qualità nazionale zootecnia, citato dall'onorevole interrogante, insieme al Sistema di qualità nazionale dedicata al tema specifico del benessere animale, rivestono sicuramente in quest'ottica un ruolo significativo. Ad oggi hanno aderito al Sistema di qualità nazionale zootecnia oltre 6.000 operatori. Siamo riusciti in questo modo ad avviare un processo di transizione verso un modello allevatoriale ancor più sostenibile e assicurare la valorizzazione delle produzioni territoriali e una corretta informazione al cittadino. Si tratta però di un processo virtuoso, ma che è su base volontaria e che intendiamo sostenere in ogni modo, dando la possibilità di verificare, specie sulla filiera delle carni, l'uso o l'abuso di prodotti come gli antibiotici. Questi sistemi saranno sempre più interconnessi grazie all'impegno fissato nella disciplina di livello europeo, che pone le etichettature nell'ottica di un quadro internazionale, che intendiamo influenzare con un'Italia sempre più autorevole in questo settore, ma dal quale non possiamo prescindere. Anzi, abbiamo contestato etichettature nazionali che invece violano le norme del libero mercato previste nei Trattati del 1957 e ancora oggi ovviamente in vigore, per garantire la massima possibilità all'interno dell'Unione europea dello scambio delle merci. Quindi, l'obiettivo credo sia comune. Riteniamo di dover lavorare in questo senso: massima trasparenza, possibilità per gli acquirenti di avere la capacità di conoscere il percorso delle merci tutte e degli animali che hanno invece un valore ancora più rilevante, essendo soggetti senzienti e capaci di provare sofferenza nel momento in cui vengono trasformati in condizioni inidonee. L'ultimo degli argomenti è quello che lei citava correttamente, e cioè la prossimità territoriale. È ovvio che questo determina vantaggi da due punti di vista: quello della sofferenza degli animali e quello delle emissioni in atmosfera dei mezzi di trasporto.

e dice di essere per la trasparenza; dall'altra, però, se ho capito bene, è contrario all'etichettatura obbligatoria. Se

Anche in Sud Tirolo abbiamo tantissimi piccoli allevatori che subiscono sempre la concorrenza delle imprese di massa, quasi imprese industriali, dove il benessere degli animali sappiamo tendere verso lo zero, ma la cui carne però costa molto di

fenomeno tanto odioso quanto incancrenito in tutto il Paese e in alcuni casi si espande anche a macchia d'olio, indistintamente su tutte le Regioni. La semplicità con cui si accede all'erogazione dei contributi comunitari e soprattutto la mancanza di controlli rigorosi rendono il sistema dei fondi europei in ambito agricolo un vero e proprio *business* per le organizzazioni criminali. Mi fa piacere vederla annuire. Vorrei ricordare, tra i tanti, il maxiprocesso dei Nebrodi, che si è concluso con condanne che, se sommate tra loro, arrivano a superare i sei secoli di carcere per reati come associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, truffa aggravata, ma anche altro. Ministro, il sistema della distribuzione dei fondi europei nel settore agricolo non funziona, e, se così non fosse, non saremmo stati costretti a leggere di un'altra

preventivi, interessando ben dieci regioni (Abruzzo, Puglia, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Campania), per un totale di 5 milioni di euro in frodi. Ministro, noi parliamo di grandi aziende che vanno ad occupare grandi aree di terreno con l'unico obiettivo di accedere a fondi comunitari, senza poi garantire l'effettiva attività di pascolo e andando anzi ad alimentare un altro odioso odioso fenomeno, quello dell'eccessivo imboschimento dei terreni. Quello che le chiediamo è in che modo intende garantire innanzitutto la sicurezza degli allevatori; in che modo intende tutelare l'economia locale dell'allevamento, controllare il corretto uso dei fondi comunitari; quali sono, in sostanza, le iniziative che lei ha messo in atto o che intende porre in essere per scongiurare e prevenire l'uso fraudolento dei fondi comunitari e porre fine agli affari sporchi della mafia dei pascoli.

che parte dalla sottolineatura di due importantissime indagini che hanno portato, dall'insediamento del nostro Governo, ad affrontare due temi quelli legati alle agromafie e alla tutela che necessitano i nostri imprenditori dell'allevamento e tutti gli altri a cui vengono sottratti soldi dalla malavita, che potrebbero andare invece a sostenere questo tipo di agricoltura. Signor Presidente, mi permetta di ringraziare, con l'occasione, la Guardia di finanza e le procure che hanno agito in maniera solerte, come fanno i nostri Carabinieri, nel controllo, per quanto possibile, di questi fenomeni che stanno diventando dilaganti anche a causa della crisi del mondo allevatoriale e di quella legata al mondo dell'agricoltura. Le indagini - come sa - sono durate due anni ed è emerso come l'associazione criminale operativa dal 2014 avrebbe simulato il possesso dei requisiti necessari per ottenere la disponibilità di terreni e di corrispondenti titoli PAC, e quindi ha beneficiato di qualcosa a cui evidentemente non aveva diritto con un'azione criminosa. Le società avevano sede - come lei sottolineava - in varie parti d'Italia. È un fenomeno che spesso avviene al Sud, ma che coinvolge attività criminose che invece hanno spesso come protagoniste persone non del Sud. ci inducono a ritenere che il sistema di prevenzione delle truffe, nonostante la dedizione e il grande impegno delle Forze dell'ordine, sia stato poco efficace. Ed è questa ragione, insieme alla necessità di affrontare le situazioni legate ai maltrattamenti degli animali, che ci ha spinti nelle ultime ore

effetto di azioni che non considero corrette, sono stati sottratti carabinieri e sono rimasti 145 uomini delle Forze dell'ordine per affrontare le agromafie e il maltrattamento degli animali, che sono un po' pochi per arrivare all'obiettivo.

era nel massimo dell'efficienza, tant'è vero che l'Europa ce lo ha contestato, in più occasioni, negli ultimi anni. Ebbene, nel decreto abbiamo eliminato un insieme di poltrone - se così vogliamo semplificare - la società SIN, che rallentava, invece che agevolare, la possibilità controlli, che ora saranno sempre più efficaci. La Commissione europea ci ha riconosciuto un efficientamento progressivo dell'Agea, perché è l'unico strumento, anche con le dotazioni di carattere tecnologico, che ci permette di incrociare i dati per essere nelle condizioni di effettuare controlli sempre più puntuali ed evitare che anche un euro finisca nelle tasche non solo della malavita, ma anche di chi non ne ha diritto. C'è una situazione paradossale, in Italia, per cui esistono allevatori che percepiscono la PAC che hanno più di centocinque anni e che riteniamo statisticamente difficile possano continuare a condurre un'attività imprenditoriale. Lavoriamo quindi in grande sintonia sintonia per affrontare problemi che non sono né di destra, né di sinistra, ma che incidono sulle tasche degli italiani e sui fondi europei, in questo caso utili a garantirci buon cibo e soprattutto tutela del territorio che viene effettuata più di ogni altra cosa dai nostri agricoltori.

prima in classifica tra i Paesi europei per frodi, e certo questo non è un primato di cui vantarsi. Ora lei mi parla di decisioni prese nelle ultime ore. io non posso essere soddisfatta da questa risposta perché questa interrogazione l'ho depositata più di un anno fa e lei, nel momento in cui è costretto a venirmi a rispondere in Aula, viene ad annunciare decisioni politiche prese nelle ultime ore: aumento del numero dei carabinieri del CUFAA, l'Agea e lo snellimento dei lavori. Vedremo Ministro, qui il meccanismo resta sempre lo stesso: intimidazioni, minacce agli allevatori locali, incendi, allevamenti di bestiame completamente rasi al suolo, animali avvelenati, grandi aziende che prendono concessioni di vaste aree

delle foreste* - Premesso che: i cambiamenti climatici in atto stanno mettendo a dura prova il comparto agricolo, che più di altri appare fortemente influenzato dalle variabili meteorologiche; Oggi vorrei trattare di un settore, quello del vino, che nel 2023 ha interessato oltre 241.000 imprese agricole del nostro Paese, con 675.000 ettari coltivati e una media di 2,80 ettari coltivati per azienda agricola. di un settore che coinvolge 33.000 aziende vinificatrici e ben 527 riconoscimenti di DOP e IGP, 77 DOCG, 332 DOC e 118 IGT. In Italia abbiamo un consumo *pro capite* di circa 37 litri annui e nell'anno 2023 i consumi totali si sono mantenuti poco al di sotto dei 22 milioni di ettolitri (meno 2 vale quasi 14 miliardi di euro, che è il 10 per cento del fatturato dell'agroalimentare italiano, ma risente della minor produzione, che è passata da circa 50 milioni di ettolitri degli ultimi tre tre anni ai 38 milioni di ettolitri prodotti nel 2023. Con riferimento al comparto vitivinicolo, la Regione Piemonte in particolare è reduce di due annate disastrose che, per via dei cambiamenti del clima, siccità estrema e delle temperature elevate, hanno segnato il quadro climatico per gli anni 2022 e 2023, influenzando senza dubbio anche l'annata che sta per arrivare. Sono piante che patiscono - lei, signor Ministro, lo sa bene - non soltanto la condizione meteorologica annuale, ma anche quella degli anni precedenti. Lo scenario descritto rappresenta una situazione di emergenza che non si è mai verificata in passato, ma che, vista la tendenza dal 2020 in poi, rischia di configurarsi come una nuova normalità con cui le aziende le aziende di settore sono costrette necessariamente a confrontarsi. Sono evidenti gli impatti a livello nazionale e i danni provocati alla viticoltura dallo stress idrico determinatosi; in ogni caso, sono recuperabili non nell'arco di un breve periodo. I viticoltori sono destinati a subire ripercussioni importanti nell'esercizio della loro attività per via di una riduzione degli introiti a fronte di un aumento dei costi di produzione. Si tratta di una situazione di grave difficoltà. Vogliamo pertanto chiederle, signor Ministro, se sia a conoscenza di queste problematiche, che probabilmente le sono state segnalate, e - dall'altra parte - quali misure intende prendere il suo Ministero su questi temi.

in maniera puntuale per la promozione dei nostri prodotti, perché l'Italia è la prima Nazione per produzione di vino ancora adesso, ma non è la prima per valore del vino esportato. Credo che il primo problema che ci dobbiamo porre è esattamente come valorizzare ancora di più quello che lei ha citato bene e che è legato ai nostri territori, alle nostre capacità di produzione e di distribuzione corretta, che ovviamente vedono il Piemonte come una Regione di eccellenza. Nelle altre Regioni possiamo ancora fare bene e soprattutto difendere quell'agricoltura che serve - e il settore vitivinicolo è protagonista in questo - a garantire la manutenzione del territorio, quella scultura del territorio che avviene con il lavoro prezioso degli agricoltori e che viene messa in discussione dalla crisi idrica che spesso - non in fase emergenziale, ma ormai spesso - da almeno un ventennio colpisce le aree del nostro Paese. Per fortuna quest'anno la situazione legata alla siccità colpisce molto di più alcune Regioni del Sud, in particolare la Sicilia, e per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene, producono un valore del vino eccezionalmente rilevante. In questi anni abbiamo avuto modo di constatare la fase non emergenziale del problema e quindi la necessità

e disperdiamo in rete quasi un litro su due. Un dato drammatico che va arginato. Stiamo spendendo inoltre tutti i fondi del PNRR utili in quest'ottica. Abbiamo portato avanti (e a termine) il rapporto con i consorzi delegati in parte alla strutturazione e lavoriamo in grande coordinamento con il MIT, con il ministro Matteo Salvini, per arrivare a

per cercare di sostenere le aziende colpite anche dalla siccità, perché ci sono tutta un'altra serie di criticità legate al mondo del vino (la peronospora prima degli altri, ma anche la flavescenza dorata) e stiamo lavorando in Europa per chiedere di condividere - perché questo l'Europa dovrebbe fare - delle azioni comuni per affrontare insieme delle emergenze che - ripeto - non fanno parte di una problematica legata a un singolo territorio, a una singola Nazione, ma derivano dagli effetti collaterali del cambiamento climatico che vanno arginati con una pianificazione di carattere più generale e con fondi idonei. vignaioli piemontesi, insieme alle altre cooperative, rappresentano ben 34 cantine di cooperative a cui sono associate oltre 5.000 aziende che rappresentano un'importante quota di produzione del settore vitivinicolo nazionale.

Infatti il rapporto tra domanda e offerta ha consentito a tutte le componenti della filiera, in passato, di avere un'equa remunerazione. Oggi però il panorama è completamente cambiato. Per garantire un futuro ai nostri agricoltori impegnati nella produzione

la diretta televisiva e ci stanno ascoltando coloro i quali seguono la televisione nazionale, la Rai, ma credo che si debba anche guardare al bicchiere mezzo pieno: i dati dicono che nei prossimi anni i consumi dovrebbero aumentare, addirittura dicono di un 10 per cento a livello di Paese fino al 2028 e addirittura a livello mondiale, del 2,1 per cento in volume e dell'8,8 per cento nel Perciò la sfida sarà proprio la capacità di sostenere e di aiutare il settore, come lei ben ha detto, attraverso la cultura dell'aiuto all'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. Siamo soddisfatti della risposta. Ringraziamo lei, Ministro, e tutto il Ministero per l'impegno. *(Applausi)*.

conosce perfettamente la situazione degli agricoltori che hanno pagato vent'anni di politica europea che ha di fatto disincentivato la produzione, pensando che si potesse smettere di produrre e acquistare le materie prime dove costavano meno, di fatto venendo meno ai principi fondanti della PAC stessa, e cioè sostenere il reddito degli agricoltori e garantire l'approvvigionamento delle materie prime. Il tutto mentre i nostri *competitor*, la Russia ad esempio diventava il primo esportatore di grano, la Cina acquisiva terreni, soprattutto in Africa, e faceva scorte di cereali, che le consentivano poi di avere uno strumento in più di geopolitica, e gli Stati Uniti giustamente sostenevano la loro economia agricola. Questa situazione, per di più, è stata acuita dalla crisi energetica prima e dal contesto internazionale di guerra poi, che di fatto hanno messo i nostri agricoltori in una posizione di forte difficoltà. Essi hanno dovuto fronteggiare poi anche le situazioni nate dal cambiamento climatico oggettivo, con il sorgere di nuove fitopatologie che hanno messo in ginocchio tanti settori dell'agricoltura e alle quali l'Europa ha dato una risposta meramente ideologica. Non ci si è concentrati sulla ricerca, sulla scienza e sulla tecnica per fronteggiare la nuova situazione, ma si è pensato di ridurre tutto ad un mero slogan, attraverso il *green deal*, che portava a considerare la sostenibilità ambientale, sbagliando anche lì, però poi nella loro declinazione, anziché la sostenibilità anche economica dei nostri operatori. È proprio in questo contesto che si è inserito il Governo

È vero, anche questo ha ereditato, signor Ministro, dai Governi che l'hanno preceduta. *(Applausi)*. Però siamo sicuri che, proprio con quell'implementazione di dotazioni dei Carabinieri e dell'ICQRF, lei saprà contrastare anche questo fenomeno. In questi diciotto mesi c'è stata una forte attenzione alle filiere, anche attraverso i bandi del PNRR, un sostegno alle nostre eccellenze, che rappresentano un modello qualitativo in tutta Europa, una forte considerazione della questione legata alle assicurazioni. In un mondo che cambia, abbiamo dovuto fronteggiare e capire con quali strumenti i nostri agricoltori potevano avere il loro reddito coperto. Ministro, contrastato quella deriva sintetica che voleva sostituire i nostri prodotti tradizionali con qualcosa di costruito in laboratorio. *(Applausi)*. Abbiamo sostenuto la ricerca attraverso le tecniche di evoluzione assistita, abbiamo studiato indennizzi per fare in modo che gli agricoltori non patissero doppiamente la crisi. E, in tutto questo periodo che ci ha preceduto, ben 5 milioni e 300.000 imprese e aziende agricole avevano chiuso in Europa. Non ultimo adesso, finalmente, un altro decreto, quello andato in Consiglio dei ministri il 6 maggio, aspettato dalle categorie produttive come acqua

Intanto voglio ringraziare il senatore Malan per aver presentato questa interrogazione e voglio ringraziare per l'illustrazione il senatore De Carlo, che ci mette più passione di altri, essendo un agricoltore arrivato in Parlamento e quindi conoscendo più di altri quanto sia importante la materia che tratta. L'atteggiamento del nostro Governo, guidato da Giorgia Meloni, da subito è stato quello di dire che per noi l'agricoltura e la pesca sono irrinunciabili in questa Nazione. a sostituirle e siamo disposti a difenderle (lo abbiamo fatto dal primo giorno) in tutte le sedi di carattere internazionale, a cominciare dall'Unione europea, nella quale probabilmente avevano dimenticato i contenuti dei Trattati di Roma e degli Accordi di Stresa dell'anno successivo, che prevedevano l'agricoltura come pilastro della garanzia di sicurezza *(Applausi)*, ma anche, dall'altro lato, della garanzia di manutenzione del territorio. La PAC era uno strumento finalizzato a questo e a nient'altro; negli ultimi anni è diventato altro e gli effetti si sono visti, purtroppo, con un decremento delle imprese agricole a livello europeo del 24 per cento e a livello italiano di oltre il 30, con punte al Sud del 45 per cento. La stessa cosa sulla pesca, con il 28 per cento di riduzione delle marinerie a livello europeo e il 40 per cento in Italia. Significa che o hanno sbagliato i Governi che ci hanno preceduto o hanno sbagliato a difendere l'Italia nei consessi internazionali, dove evidentemente le regole erano a vantaggio *(Applausi)*. L'ultimo degli atti che abbiamo proposto è il decreto-legge a cui faceva riferimento. Non basterebbero i pochi secondi che mi restano per dire che cosa abbiamo messo in campo. Abbiamo affrontato il problema del credito. Oggi abbiamo la possibilità di garantire alle imprese agricole e della pesca italiane la moratoria di un anno per i debiti che hanno contratto, se hanno superato una riduzione del 20 per cento del volume di affari. *(Applausi)*. Interveniamo con 20 milioni per ridurre il costo del denaro intervenendo sui tassi. Interveniamo altresì su una filiera che è stata messa in ginocchio dall'invasione russa dell'Ucraina e dall'invasione di grano russo dell'Italia. Per fortuna, grazie all'Italia arrivano i dazi sul grano russo e questo però deve essere anche in Italia compensato da un intervento sulle filiere del grano duro, cerealicole in particolare.

con ulteriori finanziamenti. Speriamo che in fase di conversione del decreto-legge ci sia la possibilità di ampliare ancora di più questi interventi. Abbiamo efficientato il sistema di Agricat nato quest'anno di fatto e che deve essere reso operativo. Abbiamo lavorato sul costo di produzione; si è detto durante le manifestazioni dei trattori in tutta Europa e da tempo con le associazioni agricole che era necessario garantire quelle che sono le norme che in Italia esistono sulla concorrenza sleale. E allora noi avremo un costo di produzione che verrà pubblicato e chi scende sotto quel prezzo nella contrattazione scritta diverrà

è ovviamente libero di farlo, ma se è stato indotto da anelli più forti della catena, costretto a vendere a un prezzo inferiore al costo di produzione, interverranno l'ispettorato e i nostri carabinieri per erogare le sanzioni necessarie. Abbiamo anche coinvolto i mercati con l'obbligo di segnalazione, al loro interno, di atteggiamenti contrari alle norme che abbiamo appena appena sottolineato. C'è poi la norma per l'utilizzo del suolo agricolo; si chiama suolo agricolo perché deve produrre. *(Applausi)*. La fiscalità che noi garantiamo agli agricoltori in fase ridotta è perché danno buon cibo e manutengono il territorio, non per produrre con il fotovoltaico a terra energia solare. Lo dico da Ministro che ha toccato quest'anno il *record* in termini di realizzazioni in relazione al PNRR. Abbiamo finanziato 13.500 imprese agricole che produrranno solare senza sottrarre un metro di terra un metro di terra alla coltivazione *(Applausi)*. Ci sono 1.000 modi per produrre. Abbiamo salvaguardato in questo intervento il diritto dei cittadini che avevano già fatto richiesta perché uno Stato serio mantiene gli impegni e se cambia le leggi, non danneggia quelli che hanno già presentato le domande. Abbiamo salvaguardato

oggi questo Governo interviene per risolvere il problema. Avevo accennato che non sarei riuscito a andare oltre. Ricordo ancora il commissario per la peste suina e l'intervento dell'Esercito per cercare di arrivare il prima possibile ed evitare che questa pandemia vera e propria mettesse in ginocchio la nostra economia. Per quanto

devo dichiararmi oltremodo soddisfatto, anche se naturalmente il Ministro non ha potuto, per motivi di tempo, elencare le tante misure che fanno parte di quel decreto-legge,

ideologia *green* che non consentiva incentivi alle fonti fossili. Questa Nazione, l'Italia, è l'unica che ha mantenuto lo sgravio per il gasolio agricolo, a dimostrazione di come in momenti di difficoltà bisogna essere pragmatici, cercare di

la grande missione che abbiamo è produrre di più e produrre meglio e lo si fa attraverso tanta ricerca, tanta tecnica e tanta scienza, avendo ben chiari quali sono gli obiettivi strategici della politica di questa Nazione. Oggi abbiamo un Governo che lavora sulla contingenza per lenire gli effetti disastrosi di vent'anni di governo, soprattutto europeo, ma non solo, e dall'altra parte, anche un Governo che ha una visione che ha rimesso